che in qualche maniera rappresenta tutta l'Assemblea, perché vorrei che facesse mente locale, insieme al ministro Bondi, al relatore e a tutti voi, su questo articolo 4 di cui si chiede la soppressione. Se ne chiede la soppressione perché in Italia, in cui vige il bicameralismo perfetto, se venisse approvato l'articolo 4, il Senato darebbe due ceffoni alla Camera dei deputati che su materia del tutto analoga è in dirittura d'arrivo in Commissione di merito, dacché sta concludendo l'esame del disegno di legge sullo spettacolo dal vivo. L'articolo 4 di questo decreto comporterebbe una sorta di commissariamento della Camera dei deputati

sono oltre dieci anni che le famiglie attendono da parte del Ministero un certo tipo di risposte, perché fino ad ora sono state abbastanza evasive. Peraltro, anche recentemente, gli stessi direttori di conservatorio sono stati interpellati dalle famiglie. Bisogna infatti rendersi conto che dietro le domande che fra poco le ci sono i genitori dei ragazzi che vorrebbero una certa sicurezza riguardo al percorso formativo dei loro figli. Come stavo dicendo, gli stessi direttori di conservatorio, anche recentemente interpellati, nonostante siano stati ripetutamente convocati presso il Ministero a Roma per ottenere dei chiarimenti sui percorsi didattici, danno delle risposte opposte tra loro. Se mi permette, nessuno ha ben capito la direzione che si intende intraprendere. Gli studenti hanno posto delle domande serie: i privatisti potranno terminare il loro percorso di studi? Alcuni danno delle risposte affermative, mentre altri sostengono che non sarà possibile. Qualcuno sostiene che si devono iscrivere subito al conservatorio per poter accedere immediatamente ai corsi con il nuovo ordinamento; qualcun'altro ancora sostiene che bisogna aspettare le successive scadenze che verranno poste dal Ministero. In questo ultimo anno scolastico - altra domanda - sarà possibile terminare gli studi con il vecchio ordinamento, stante che ancora non sono state diramate direttive precise? Il privatista potrà dare gli esami intermedi nei corsi di studio? Signor Ministro, con questo emendamento si tenta di dare una risposta abbastanza celere perché i tempi per iscriversi al conservatorio con il nuovo ordinamento sarebbero già scaduti il 30 aprile. Capisce bene che tanti di questi studenti, tante di queste famiglie, sono nel guado: non sanno da che parte stare, non sanno come comportarsi, e certamente non ammettere questo emendamento, come ha suggerito il relatore, o ancor peggio sollecitarne il ritiro, non depone certamente a favore dell'attenzione che questi giovani studenti di musica si aspettano.

tratta infatti di un argomento sul quale anch'io ho interpellato il Ministro con molte interrogazioni formali senza avere risposte. È questo un argomento che riguarda moltissimi giovani. Mi rendo conto che il ministro Bondi e il relatore possono dire che è materia che dovrebbe essere altrove, anche questa mattina abbiamo ricordato che esiste una collegialità del Governo: se un Ministro fa la riforma della scuola secondaria un altro collega forse deve saperlo e in quella maniera integrare le forze. Non avendo potuto avere avere chiarimenti anche su coloro che saranno gli eventuali insegnanti, a me sembra che questo emendamento sia in questa sede opportunamente collocato e, se i colleghi hanno colto le argomentazioni del collega Stiffoni, vale la pena che lo votino.

non può parlare nessuno e tantomeno il relatore. Lei deve far votare adesso e togliere la parola al relatore.

ai quali quando il Presidente di un Gruppo ha chiesto la parola, anche in questa fase, gli è stata data. È stata data tante volte alla senatrice Finocchiaro, e si deve dar atto

relatore avrebbe chiesto la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento, con un impegno morale a far entrare tale norma all'interno di un disegno di legge

di chiedere ai colleghi della Lega, e innanzitutto al senatore Stiffoni, di votare contro questo emendamento, dal momento che siamo in fase di votazione, fermo restando l'impegno politico e morale a fare ciò che si sarebbe fatto attraverso la trasformazione in un ordine del giorno.

Onorevoli senatori, non posso non condividere quello che ha detto poc'anzi il senatore Gaetano Quagliariello.

nelle competenze del Ministero della pubblica istruzione. Ritengo quindi doveroso, anche per rispetto al Ministro della pubblica istruzione,

Senatore Legnini, se non passano i 20 minuti dal preavviso non posso dichiarare aperta la votazione, e quindi non siamo in votazione. Comunque, la Presidenza fa presente che ci sono precedenti consolidati.

dei lavori, ma la disattenzione nei confronti della regola era già iniziata ed è proseguita comodamente, come se stessimo chiacchierando in fase di illustrazione dell'emendamento e prima della votazione.

il problema non è più procedurale, tant'è vero che ha invitato i colleghi della Lega Nord a votare contro l'emendamento 4.300, riconoscendo che siamo in una fase del procedimento in cui non si può revocare la votazione. Pertanto, se questo emendamento viene bocciato, viene bocciato: ci sarà eventualmente poi un ordine del giorno o un'altra iniziativa, ma credo che forzare la mano in questa fase - e devo dare atto ai colleghi della maggioranza che non lo hanno chiesto e non lo hanno fatto - significherebbe creare un precedente che poi diventerebbe antipatico

Signor Presidente, si stanno facendo tante polemiche su una questione che si poteva invece risolvere in maniera diversa.

Presidente, poco fa Stiffoni mi ha concesso l'onore di sottoscrivere il suo emendamento. Pertanto, sono nella condizione di non rinunciare all'emendamento e di non accettare la sua trasformazione in ordine del giorno.

Pertanto, nel caso di specie, quando il titolare dell'emendamento ne chiede la trasformazione in ordine del giorno non vale la seconda sottoscrizione. Senatore Stiffoni, insiste per la trasformazione in ordine del giorno o chiede il voto dell'emendamento

signor Presidente, la pregherei di suggerire alla collega Garavaglia che forse è il caso di avere un ordine del giorno che - visto l'impegno assunto dal ministro Bondi - sarà pregnante anche per il futuro esito

mi auguro che il Senato rispetti quelle poche regole che sappiamo esservi e che non possono essere cambiate come se si giocasse una partita al gioco delle tre carte. Se sono esperti dall'altra parte, noi non siamo completamente distratti. Siamo in fase di votazione. Bisogna votare. Poi,

non l'abbiamo prodotto noi questo imbarazzo. Rispettiamo, dunque, le regole e vedremo; vorrà dire che la Lega Nord, che ha presentato l'emendamento, voterà contro. Però, la coerenza e le regole sono la stessa cosa. Noi le dobbiamo portare avanti.

Presidente, noi abbiamo la fortuna di trovarci in una fattispecie che il nostro Regolamento definisce in modo lineare.

non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso».

la votazione deve essere conclusa. Poi torna naturalmente nella disponibilità del Presidente concedere la parola per gli argomenti per i quali verrà richiesta. La ringrazio molto se vorrà dare esecuzione al disposto dell'articolo 110 del nostro Regolamento.

Per quanto riguarda il secondo problema dell'ordine del giorno, senatore Stiffoni, esso è già stato posto all'attenzione alla Presidenza. Senatrice Garavaglia, il Regolamento che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati. Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiederne la votazione. *(Commenti Ciò premesso, senatore Stiffoni, o lei ritira la sua richiesta di trasformazione in ordine del giorno e si vota l'emendamento, e noi andiamo avanti nei lavori, oppure noi dobbiamo prendere atto che ha ritirato l'emendamento. *(Commenti

entro nel merito dell'emendamento e, quindi, della proposta di trasformazione in ordine del giorno fatta dal senatore Asciutti. Il senatore Asciutti sa bene quanto me, avendo concorso insieme alla stesura

provvedimento, da quando è stato approvato, con una votazione trasversale che ha visto il voto da Alleanza Nazionale fino all'estrema Rifondazione Comunista, non ha trovato il modo di viaggiare in questo Paese e di avere piena attuazione, in quanto i regolamenti sono stati regolarmente boicottati.

Questo signore si è permesso fino ad oggi - lo sanno tutti, caro Ministro - di ostacolare la riforma che abbiamo votato in questo Parlamento, che è legge dello Stato e che non riesce ad espletare tutte le sue indicazioni e funzioni perché c'è la volontà, da parte del Governo, di frenarla. Caro collega Stiffoni, non ti fidare, perché l'ordine del giorno non serve a nessuno:

che equipara i titoli di studio che essi rilasciano a livello europeo come titoli di studio universitari. Allora, in questo Stato si fanno leggi che poi si disattendono perché i funzionari o i dirigenti remano contro? O c'è la volontà di un Governo di consentire ai funzionari di remare contro penalizzando un'intera area, del comparto musicale e artistico italiano? Non si può più consentire ciò. Non farti prendere in giro, collega Stiffoni: non è da te, né dalla Lega. Non fatevi prendere in giro, e non prendiamoci in giro: l'ordine del giorno non serve a nessuno.

Secondo gli Uffici risolutiva. si determinerebbe un precedente molto grave, non starei qui ad insistere. Non devo essere io a dirle che il procedimento della votazione si apre con l'indizione della votazione, che si può fare dal primo minuto

il procedimento, che è già iniziato, si sospende, in attesa che passino i 20 minuti. Questo è chiarissimo. L'argomento che lei pone invocando una prassi - che non so dove abbia rinvenuto - è *contra* Regolamento e non può essere accettato in alcun modo. Far fare ingresso a questo argomento nella conduzione dell'Aula vuol dire che da questo momento in poi possiamo fare quello che vogliamo: si apre la richiesta, si sospende, poi si tratta, si discute, si ritira e poi si trasforma. Lei ha un modo molto semplice per risolvere il problema: azzerare tutte le chiacchiere fatte dal punto di vista dell'incidenza delle decisioni e far votare. Il Gruppo della Lega, che ha peraltro detto che voterà contro il suo emendamento, se ne assuma la responsabilità. Il problema è risolto. Se lei non fa questo, Presidente, mi

consideravo e continuo a considerare questa materia importantissima. Anche nel mio primo intervento ho detto che non era proprio il posto giusto, ma c'è una collegialità nel Governo: non sarà un modo per ferire le competenze reciproche del ministro Bondi e del ministro Gelmini. Credo che questa norma, se fosse approvata, renderebbe un grande servizio

di tutti i successivi emendamenti a ritirarli, in quanto c'è la soppressione dell'intero articolo 5, già approvato in sede di Commissione.

sbagliato nei contenuti e nel metodo: nei contenuti, perché trasforma, altera e restringe la missione di Cinecittà; nel metodo perché interviene pesantemente per decreto nel settore cinematografico,

L'ordine del giorno. G7.100 non è inerente alla materia, quindi inviterei il

di un istituto che è al momento commissariato, su cui pesa un'indagine piuttosto rilevante della magistratura; non stiamo cioè parlando di varie ed eventuali, ma di uno dei passaggi più delicati. Fummo noi i primi a dire - il Ministro e il Sottosegretario lo ricorderanno - che questo è l'unico punto che merita un'effettiva urgenza: si stralci questo argomento e facciamo di esso un punto anche unitario.

che rischia di vanificare lo sforzo di mantenere in vita l'istituto mutualistico degli artisti.

non sono in discussione né il diritto degli artisti a vedersi riconosciuti i loro trattamenti economici,

Dico questo perché l'IMAIE, che è appunto l'istituto mutualistico preposto alla tutela dei diritti degli artisti, interpreti, esecutori che ridistribuisce agli aventi diritto i soldi provenienti dai passaggi nelle televisioni, e dunque anche nelle televisioni Mediaset (ecco perché ho parlato di conflitto di interessi del cavaliere Berlusconi), si vorrebbe sostanzialmente metterlo sotto la vigilanza del Governo - questa è l'anomalia - quindi della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni culturali e del Ministero del lavoro. La storia dell'IMAIE è piuttosto lunga e non la ripercorro, anche se sinteticamente ricordo che l'Istituto ha avuto una vita molto travagliata. In ultimo, l'anno scorso il prefetto di Roma aveva sostanzialmente commissariato (non è il termine tecnico giusto, ma lo uso tanto per capirci) l'IMAIE per assoluta incapacità di raggiungere gli obiettivi statutari, perché da una relazione dei revisori dei conti era emersa una grave situazione finanziaria e, soprattutto, una incapacità dell'ente non non solo di ottenere i fondi che avrebbero dovuto essere erogati dalle televisioni, dunque il pagamento dei diritti, ma tantomeno di redistribuirli. Soprattutto, era emerso che nel 2007 vi erano 120 milioni di euro da redistribuire e dopo due anni questi soldi, pur non distribuiti a nessuno,

è stato emanato il decreto d'urgenza che ha introdotto la norma sull'IMAIE che, tra l'altro, non è assolutamente conferente rispetto ad un riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche. Dunque, è legittimo il sospetto che questa norma si sia voluta introdurre *ad hoc* per non arrivare alla decisione del TAR. Il Ministro anche su questa questione sembra voler andare avanti a tutti i costi, nonostante le sollecitazioni anche delle opposizioni di stralciare la materia per arrivare ad una definizione che - lo ripeto - tuteli (questo è l'interesse dell'Italia dei Valori) i lavoratori innanzitutto, ma anche e soprattutto i diritti degli artisti. Ma, con prepotenza questo non si è voluto. Ed allora noi crediamo che per come, fra l'altro, è strutturata questa norma si potrebbe arrivare a difficoltà nell'accertamento delle eventuali (perché ad oggi non esistono

riconosce anche, lo dico da esponente del Nord, il ruolo dei precursori. Lasciatemi citare in particolare, perché c'è una bellissima zona che li ricorda, il ruolo del movimento

determina un onere che si copre con una copertura permanente di aumento dell'accisa sui tabacchi, per una festività nazionale in più che nel testo dell'emendamento 7.0.70, di cui questo è un subemendamento, è stabilita solo nel giorno 17 marzo 2011.

ho visto distratto il senatore Legnini mentre parlavano il senatore Morando e gli altri senatori, così come ho visto distratto il senatore Zanda. pare però di capire che, se si è in votazione in un certo modo, allora ci si appella a quel Regolamento al quale ha fatto riferimento con la mano in tasca e l'indice vindice il senatore Legnini; se invece è da curare e da modificare un evidente errore di questa minoranza, allora tutto va bene. *(Applausi dal Gruppo* *PdL).* Vorrei soltanto sapere come funziona: non sto facendo critiche a nessuno, tanto meno al signor Presidente che mi ascolta. La mia è soltanto una richiesta di informazioni:

intervengo per dichiarazione di voto a titolo personale, poiché ritengo che inserire nel calendario un'ulteriore festa nazionale - pur trattandosi dell'unità del nostro Paese

saccheggiare la voce delle accise, senza toccare mai il fondo, finisce per comprimere e, soprattutto, per rendere impossibile la vita a circa 200.000 industrie

data dell'anniversario dell'Unità d'Italia debba coincidere con una giornata di astensione dal lavoro. Non entra nel merito perché non tocca a questa normativa e nessuno di noi l'ha pensato.

a cui il Senato ha molto contribuito, e di cui va dato atto a tutte le massime cariche dello Stato, di uno studio molto approfondito e di una grande riconoscenza

il 17 marzo 2012 sparirà dal calendario mi sembra, anche rispetto alle tradizione degli altri Paesi europei a cui facciamo riferimento, un dato

con l'astensione della Lega riguardava esclusivamente una giornata, quella in cui

l'emendamento 7.0.500, che riguarda la Fondazione dell'orchestra Verdi di Milano. Con questo emendamento avviava finalmente la presa in carico di un impegno che ha protocolli che riguardano due Governi precedenti; finalmente si concretizzava questo impegno per una grande istituzione culturale milanese che si è fatta da sola.

come orchestra sinfonica è una delle realtà più importanti del Paese - senza mai ricevere una lira dalle istituzioni pubbliche. Adesso si trova in difficoltà e c'era l'impegno di tutti (Comune, Provincia, Regioni e Stato) a darle una mano.

è solo per tre anni; bisognava semplicemente scrivere: «a partire dal 2010» anche per quello che riguarda la copertura. Così avevamo concordato, ma poi anche se da me non condivisa - di ritirare l'emendamento: è una decisione politica presa dal relatore, immagino d'accordo con il Governo, che con il parere contrario della Commissione bilancio obiettivamente non c'entra niente. PRESIDENTE. Riprendiamo l'espressione

contrarietà alla soppressione dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, sui servizi aggiuntivi. Riteniamo infatti che tramite i servizi aggiuntivi possa dare ai nostri musei e siti archeologici un migliore servizio e una maggiore concorrenzialità; crediamo che l'introduzione di questo articolo porti invece a privilegiare le grandi multinazionali della cultura che non permetteranno il libero svolgersi delle competizioni all'interno di questi siti. Sosteniamo pertanto con forza l'emendamento 8.27. Signor Presidente, parliamo di una norma, ancorché apparentemente marginale, molto importante. Mi rivolgo al Ministro,

Di che cosa si tratta e in che modo noi, nella situazione del territorio italiano, intendiamo operare per quanto riguarda i servizi aggiuntivi? È evidente che stiamo parlando di una materia che, come sappiamo, fu introdotta dal compianto collega Ronchey, che per la prima volta portò nelle istituzioni culturali italiane i cosiddetti servizi aggiuntivi, ovvero la possibilità che privati potessero portare *bookshop*, bar, ristorazione ed altre attività private integrate con il servizio erogato dal pubblico. Come si deve svolgere questo servizio? Pensate a musei di piccole realtà, dove non vi è la massa critica per aprire un *bookshop*; ma pensate anche alla qualità complessiva dell'offerta. La proposta di abrogazione che avanza il Governo, ministro Bondi, sostanzialmente prefigura lo "spezzatino" ovvero che ciascuno si debba occupare del suo comparto. Chi fa le pulizie crei il cartello delle pulizie, chi si occupa dei *bookshop*, della vendita di libri e prodotti culturali, faccia il cartello dei *bookshop*, chi si occupa della ristorazione o dei bar La proposta precedente, che so bene, Ministro, è stata contrastata anche in nome del desiderio di creare degli spezzatini e dunque di diffondere non la qualità dell'offerta, non una capacità competitiva con i grandi musei internazionali, ma delle situazioni parcellizzate e non necessariamente, colleghi, efficienti e fruttuose per il pubblico, è stata combattuta in nome del desiderio di non creare degli aggregati competitivi in grado di fornire dei servizi sul grande mercato che - voglio ricordare -noi abbiamo interesse di formare, perché in Italia ci sono 4000 musei. Non abbiamo soltanto i circa 400 luoghi-musei e luoghi archeologici dello Stato; abbiamo migliaia di musei dei Comuni, musei diocesani, musei privati, che hanno bisogno di avere l'interlocuzione di soggetti in grado di produrre un'economia di scala ed una qualità dell'offerta verso il grande pubblico, quando questo viene fatto in modo integrato. Prendiamo le Scuderie del Quirinale, struttura che io ebbi l'onore di costruire, assieme al collega Zanda, in occasione del del Giubileo: era infatti una struttura abbandonata. L'attuale amministrazione ha salutato una grande mostra, quella del Caravaggio, con più di mezzo milione di visitatori, con grande introiti per la componente di *bookshop*, di ristorazione e dei servizi connessi, perché è un sistema nel quale è possibile il collegamento con altre istituzioni culturali. Lo spezzatino, signor Ministro, non è convincente. Le chiedo di riflettere attentamente, perché vi richiameremo su questo ad una verifica del risultato dello spezzatino nel momento in cui incentivate i cartelli e - aggiungo - non fate altro che lamentarvi del fatto che le sovrintendenze territoriali

ad un livello più alto, basato sulla qualità, sulla fornitura di servizi che costringono con associazioni temporanee di impresa le diverse aziende specializzate (chi nelle pubblicazioni, chi nella pulizia, chi nella ristorazione) a fornire un'offerta complessiva e qualificata, voi caricate sulla sovrintendenza di Reggio Calabria la gara per la pulizia, per il bar, per il *bookshop*. Si scoprirà che la gara per il *bookshop* del museo di Locri va deserta, perché è molto difficile creare la massa critica per farla funzionare. È questa la direzione di un'economia sociale di mercato e di una capacità di portare nelle politiche per la cultura quella integrazione dei servizi degna del nostro grande patrimonio e della necessità di dare un'offerta adeguata al grande pubblico, in un momento di crisi del turismo e delle risorse pubbliche per la cultura, attirando risorse private? Mi perdonerà, Ministro, se sono appassionato sulla questione, ma come lei sa sono materie di cui anche io personalmente mi sono occupato nella mia prima esperienza di sindaco e poi nei 20 mesi in cui sono stato Ministro dei beni culturali, anche cercando di integrare questa opportunità con quella del turismo.

- liberale, rivolta alle condizioni della concorrenza, ad un'economia di scala nel settore della cultura ed al miglioramento dei servizi per i milioni di visitatori potenziali nei musei e nelle aree archeologiche, i quali, quando nasceranno queste associazioni di impresa, potranno vederle integrate con i musei locali, con il circuito dei musei civici e con tutte quelle strutture (laiche, religiose e private) che formano la grande ricchezza del patrimonio culturale del nostro territorio. Ecco perché

riprende la prima parte dell'emendamento 3.138, mi ritengo soddisfatto, perché in esso viene ricompresa

esaminando, di fatto, crea dei problemi di carattere sociale gravi nei confronti di un numero abbastanza circoscritto di soggetti, che sono artisti di altissimo livello e di altissimo pregio (stiamo parlando di qualche centinaio di ballerini), perché saranno obbligati, il giorno dopo la definizione dell'*iter* di questa conversione, ad andare in pensione. Cosa chiediamo, invece, con questo emendamento, signor Ministro? Che ci sia la possibilità di prevedere un ammortizzatore, che non costa nulla ma addirittura crea vantaggi per l'istituto, quello di poter avere in cinque anni la possibilità di uscire fermo restando comunque che non si possa andare oltre i 47 anni per le donne e oltre i 52 anni per gli uomini. Non capisco il motivo per il quale non si voglia raccogliere questa esigenza, questa istanza decisione è in controtendenza anche per quel che riguarda la gestione da un punto di vista economico dei sistemi pensionistici. Ecco il motivo per il quale chiedo al signor Ministro e al signor relatore

di riflettere insieme sullo stesso. Fare questo scelta significa condannare delle persone ad una pensione forzata minima che, in alcuni casi, non supererà i 700, 800 euro al mese.

Vi invito a riflettere e invito i colleghi a valutare con attenzione, anche in un momento di orgoglio di quest'Aula, se, di fronte ad un tema che non produce aumenti economici, che ha una forte valenza sociale e che richiede rispetto nei confronti di persone che hanno dedicato e dedicano una vita all'arte, quest'Aula può avere la volontà di decidere. E qualora il signor relatore

onorevoli senatori, siccome questo tema è particolarmente delicato e ci abbiamo lavorato a lungo, ci è sembrato

e vorrei aggiungere, perché probabilmente nella stesura del testo è venuta meno, una modifica all'emendamento: questo per un motivo di correttezza.

Presidente, così, a prima vista, sembrerebbe non comportare profili di onerosità.

di anni 47 per le donne e di anni 52 per gli uomini». Questa è la dizione esatta che soddisfa sia i requisiti della Commissione bilancio che i requisiti di merito proposti dal senatore Tofani.

*(PdL)*. Dico al senatore Asciutti, ai colleghi e ai membri del Governo che per me questa soluzione va bene, mi sembra valida, però «rinnovabile annualmente» cosa significa più se è solo l'arco di due anni ad essere interessato da questa opzione?

questo emendamento nella sua versione originaria, il passaggio da cinque anni a due anni non è irrilevante. È evidente che due anni sono meglio di zero, però si era parlato di almeno tre anni. L'opinione del nostro Gruppo è di astenersi su questo emendamento.

il provvedimento che oggi è prossimo al voto finale del Senato non è l'attesa (e ormai per noi indispensabile) riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche che dovrebbe, a distanza di più di dieci anni dal decreto legislativo n. 367 del 1996, ripensare l'intero comparto alla luce di tutto quello che l'esperienza di questi anni e l'analisi dello stato delle fondazioni ha messo in luce. Si tratta, piuttosto, di un provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, si limita a tagliare, in maniera indiscriminata e in assenza di una vera strategia riformatrice, i costi del personale, intervenendo sui contratti in essere in una maniera che, che, per alcuni versi, appare anche a noi incostituzionale. L'impostazione generale del decreto tende, infatti, a identificare nel costo del personale il principale, se non unico, elemento di spreco del sistema da correggere attraverso tagli che non sono frutto di una corretta revisione degli istituti contrattuali, ma solo un intervento acritico e centralista di riduzione delle parti variabili dei salari. Ora, è di tutta evidenza come questa impostazione, signor Presidente, che identifica nel costo del personale l'unico parametro su cui intervenire, è in palese contraddizione con il fatto che, nel caso specifico dei teatri dell'opera (e comunque nel settore più ampio dello spettacolo dal vivo), il personale rappresenta l'elemento più importante e, a nostro avviso, imprescindibile per costruire il prodotto teatrale: l'opera lirica, i concerti sinfonici, i balletti, gli spettacoli di prosa non potrebbero aver luogo senza professori d'orchestra, artisti del coro, ballerini, tecnici, macchinisti, costruttori, che costituiscono proprio quella voce di costo sulla quale il Governo intende intervenire con il decreto oggi in discussione. Questo insieme di professionisti dello spettacolo è un pezzo del patrimonio culturale del nostro Paese. Senza di essi il grande melodramma, che rappresenta da sempre uno dei prodotti più importanti dell'Italia nel mondo, non potrebbe ogni sera essere messo in scena in tutto il nostro Paese. E, alla fine, l'Italia sarebbe più povera di quello che già è per effetto delle politiche culturali miopi del Governo. Poiché non è immaginabile che il Governo intenda mettere ulteriormente in crisi un settore così centrale per l'identità e lo sviluppo del nostro Paese, si deve dedurre la palese volontà del Governo di utilizzare lo strumento di questo decreto per creare le condizioni per obbligare le parti a portare a conclusione la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro entro un breve termine, pena l'attivazione di misure gravemente lesive dei diritti acquisiti dai lavoratori, come il previsto taglio della parte economica degli integrativi aziendali. Mettiamo subito in chiaro che anche noi pensiamo che sia molto grave che il contratto sia scaduto da tanti anni e che le parti non siano riuscite a firmare quello nuovo. Anche noi pensiamo che il contratto debba essere rinnovato in tempi brevi e che con il rinnovo vadano rinegoziati molti istituti che oggi appaiono anacronistici, che hanno creato le premesse per situazioni di spreco delle risorse e anche, in qualche caso, hanno garantito privilegi da eliminare. Ma non può certo essere ipotizzabile che per ottenere il rinnovo del contratto scaduto da troppi anni si ricorra a un metodo ricattatorio minacciando di intervenire per decreto sulla contrattazione. Vi è poi da fare una riflessione sulla scelta di affidare all'ARAN la responsabilità della contrattazione. Qui va sciolto un equivoco ormai insostenibile e risolta un'ambiguità che il Governo da alcuni anni sta pericolosamente alimentando, determinando confusione e ulteriore incertezza in questo mondo. da una parte si continua a invocare una dimensione privatistica per i grandi teatri d'opera, che dovrebbero attrarre sempre di più risorse private, che dovrebbero muoversi in un contesto di efficienza gestionale tipico dell'impresa privata, che dovrebbero garantire il ricorso a modalità privatistiche di gestione dei rapporti contrattuali, dall'altra parte si continuano a proporre interventi che riportano ad una concezione statalista con un progressivo rientro dei teatri nell'alveo della funzione pubblica che certamente stride fortemente con la loro natura privatistica. Mi riferisco ormai patologico al commissariamento, alle norme che vincolano tutte le azioni relative alle politiche di bilancio e a quelle di reperimento del personale a un controllo asfissiante da parte del Ministero. Signor Ministro, almeno in dichiarazione di voto non mi pare interessato. Mi riferisco alla totale mancanza di autonomia gestionale che dovrebbe caratterizzare in maniera virtuosa queste istituzioni culturali che dal 1996 hanno iniziato un percorso di privatizzazione che semmai va completato ma non certamente affossato con il loro rientro nella sfera della funzione pubblica. Ci dica con chiarezza il Governo - signor Ministro, ancora una volta: ci ascolti per favore! - se ritiene le fondazioni liriche organismi privati o pubblici e si comporti poi di conseguenza. Noi pensiamo che il percorso aperto dal decreto legislativo Veltroni vada completato, che vadano create le condizioni garantite dallo Stato minime di sostenibilità. Ci pare che il Governo vada in una direzione assai opposta, che intenda più che garantirne la sostenibilità assicurarsi un sistema di controllo su di esse. E questo è, a nostro parere, un errore molto grave. Qui serve davvero una riforma di settore. Ma non è attraverso un decreto taglia-spese che si riforma un settore così delicato e così complesso che rappresenta l'ossatura culturale del territorio, che rappresenta uno dei più forti e concreti elementi identitari del nostro Paese. Né si può qui tacere della volontà manifesta nel decreto di indurre forme di precarizzazione del lavoro anche in un campo così delicato come quello della cultura. Il blocco del *turnover*, il ricorso a contratti a tempo per via del blocco delle assunzioni, il limite nella possibilità di assumere anche a tempo determinato sono misure che avranno, se approvate, un effetto devastante sull'intero sistema e, in particolare, sui complessi artistici che rappresentano l'asse portante dei nostri teatri d'opera. Forse, signor Ministro, avrebbe fatto bene ad ascoltare il grido che si è levato dai grandi artisti che lavorano nei nostri teatri e che, certo, meglio di tutti noi conoscono la specificità del loro lavoro e la specificità del lavoro nelle nostre istituzioni musicali. Avrebbe fatto bene, signor Ministro, almeno ad ascoltare Carla Fracci, Zubin Mehta, Luca Ronconi. Perché, certo, prima di mettere mano a un settore così strategico per la crescita del Paese e così complesso e particolare, sarebbe stato utile sentire oltre agli operatori del settore anche i grandi artisti, il cui parere disinteressato avrebbe potuto illuminare e orientare le scelte del Governo. Cosa dicono da mesi questi grandi artisti? Signor Ministro, dicono che è importante la stabilità, è importante il far musica insieme, è importante crescere insieme come gruppo. Dicono che è importante selezionare i migliori talenti attraverso concorsi pubblici internazionali e poi mantenere una dimensione di competitività internazionale garantendo stabilità del rapporto di lavoro. Con la precarietà si perdono i migliori talenti e il Paese ancora una volta si impoverisce. È ancora più preoccupante il fatto che dalla lettura del decreto emerga la volontà del Governo di introdurre elementi di riforma del sistema attraverso successivi regolamenti da emanare. È paradossale, signor Ministro, che il Governo pensi di procedere a riformare il settore attraverso regolamenti e preveda di tagliare le spese attraverso un decreto-legge. Anche perché gli elementi di preoccupazione, a questo riguardo, sono tanti. In primo luogo va sottolineato come la risposta che il Governo immagina di dare all'esigenza ormai sentita da tutte le parti coinvolte di riformare il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, piuttosto che passare da un condiviso percorso legislativo parlamentare, possa realizzarsi attraverso l'adozione di questi regolamenti. Il sistema ha necessità di una riforma di settore profonda che, in prima istanza, costituisca le condizioni affinché il più innovativo dei principi previsti dal decreto legislativo n. Nonostante le tante promesse, infatti, il Governo non ha mai lavorato seriamente su un *corpus* di norme che fornisse ai privati quegli incentivi fiscali, sul modello dei Paesi del mondo anglosassone, che rendono vantaggioso per il privato il finanziamento della cultura. Non c'è occasione in cui il Governo non abbia riconosciuto come imprescindibile un intervento di questo tipo, non c'è stato convegno, seminario, dibattito in cui non si è affermata la necessità di dotare il nostro sistema di quegli incentivi che sono alla base del finanziamento privato

Anche su questo, il Governo sia chiaro una volta per tutte e poi sia conseguente: se, come è giusto, la strada è quella di incentivare i privati, il Governo vari subito le norme di defiscalizzazione indispensabili; se, invece, non ha la forza di predisporre tali norme, garantisca all'intero comparto dello spettacolo le risorse necessarie per vivere dignitosamente e per svolgere la missione per la quale esiste. E siamo così al problema principale e irrisolto: quello delle risorse finanziarie. Lo ha detto in Commissione nei suoi interventi anche il sottosegretario Giro: le risorse per lo spettacolo sono sostanzialmente invariate dal 2003 ad oggi; il che vuol dire che, tenendo conto, del tasso di inflazione, lo stanziamento ha subito una riduzione di fatto di circa il 30 per cento diventando assolutamente sempre più inadeguato rispetto alle esigenze del settore. È proprio questo quello che da anni si lamenta da parte di tutti gli operatori del settore. D'altra parte, la sofferenza del comparto è notevole soprattutto in relazione alla persistente incertezza - lo vogliamo dire con molta chiarezza - delle risorse su cui si potrà contare nei prossimi anni e al gravissimo ritardo con cui ancora vengono erogate, costringendo le fondazioni all'indebitamento e al pagamento di notevoli cifre per interessi passivi. È indispensabile che qualunque intervento da parte del Governo si ponga l'obiettivo prioritario di dare certezza almeno triennale all'intero comparto delle fondazioni: signor Ministro, non solo a quelle fondazioni cui il Governo avrebbe intenzione di conferire uno *status* di autonomia rispetto alle altre. Allo stesso tempo va assicurato un sistema di di anticipazioni ad inizio di anno che evitino il ricorso all'indebitamento. Così come è ovvio che lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo deve essere riportato a livelli compatibili con la sostenibilità dell'intero comparto. Siamo molto al di sotto del minimo indispensabile per il 2010. Il Ministro sa bene che, se le risorse previste per il 2011 non dovessero essere reintegrate,

non c'è più tempo da perdere. Ci vogliono più risorse per il settore, deve essere garantito il finanziamento triennale per tutti e le risorse disponibili vanno erogate in anticipo, interrompendo la spirale dell'indebitamento di cui stiamo parlando. Signor Ministro, ancora una mortificazione del lavoro della Commissione istruzione, che con una risoluzione approvata l'anno scorso tracciava le linee guida di una vera riforma. Noi siamo convinti che dietro una riforma ci debba essere un'idea: qui non c'è nessuna idea. Ancora oggi, questa mattina in Aula, un'altra mortificazione rispetto al lavoro della Commissione istruzione: perché non si è impegnato, signor Ministro, a trovare le risorse rispetto al 5

colleghi, il nostro Gruppo condivide l'esigenza di riforma del settore lirico-sinfonico, emersa in più occasioni nel corso dei dibattiti dedicati a questo tema nella 7a Commissione, di cui esemplificazione è proprio l'approvazione sull'argomento di una risoluzione unanime nel marzo 2009 dai cui contenuti sarebbe stato, a nostro avviso naturalmente, più opportuno partire. Siamo infatti consapevoli che continuando di questo passo non andremo avanti se non verso il collasso del comparto. Tuttavia riteniamo che questo provvedimento non sia adeguato per rispondere alle esigenze di un settore così in crisi e per far fronte effettivamente alla emergenza in cui esso versa. Non lo è, a nostro avviso, né nel merito né per il metodo che avete voluto adottare. Riteniamo in primo luogo inappropriato ricorrere alla decretazione d'urgenza: un disegno di legge sarebbe stata la forma più consona, soprattutto perché con questo decreto si incide molto marginalmente. Non si affronta, infatti, il tema più importante, quello della *governance*, e tanto meno quello della maggiore responsabilizzazione degli enti, onde far corrispondere le spese alle effettive risorse disponibili, ma si attribuisce, di fatto, una ennesima delega in bianco al Governo per il riassetto del settore e - cosa molto strana - senza indicare peraltro un binario culturale, oltre che tecnico, in cui una delega deve naturalmente muoversi. Deleghe in bianco non se ne danno mai. Non ci convince inoltre il merito. Non ci convince inoltre il merito. L'unico aspetto su cui il decreto-legge si sofferma, infatti, è il costo del personale, cosa sacrosanta, per carità, che però viene affrontata in maniera molto impropria e per certi versi addirittura, come è stato rilevato, illegittima. La legge Veltroni del 1996 - lo ribadisco senza nessun rimpianto - ha fallito, e gli effetti di tale fallimento sono sotto gli occhi di tutti. Non è affatto pleonastico ricordare come per il nostro Paese l'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche sia di enorme importanza, perché profondamente significativa è la cultura sinfonica dell'Italia, che è tra le prime del mondo, nonché di lunga e autorevolissima tradizione. Caro Ministro, se si parla italiano in alcuni angoli sparuti del mondo spesso lo dobbiamo anche, se non esclusivamente, alla nostra tradizione lirico‑sinfonica: basta andare in Giappone per verificarlo. Per la sua peculiarità e ricchezza, questo patrimonio merita un'attenzione particolare e una disciplina che non è paragonabile a quella di altri Paesi proprio in ragione della sua eccezionalità. Nessuno nega (come noi non abbiamo negato) la necessità di una razionalizzazione dei costi, e soprattutto non si può non riconoscere il fallimento ‑ come qui è stato detto ‑ della gestione da parte dei sovrintendenti, vista la situazione drammatica del settore. Ma non è penalizzando i lavoratori che la situazione potrà essere sanata, in particolare alla luce del difficile periodo storico, quanto piuttosto responsabilizzando la gestione delle fondazioni sino ad oggi troppo disinvolta e poco consapevole, nonché creando opportune sinergie finalizzate alla riduzione dei costi e soprattutto delle produzioni. È necessario peraltro applicare al settore dei criteri imprenditoriali - così com'è si è tentato di fare - che responsabilizzino le figure manageriali rispetto alle scelte da fare sotto l'egida di controlli più stringenti ed efficaci rispetto a quanto fatto dall'attuale dirigenza. Occorre perciò puntare il dito sulla responsabilizzazione e la razionalizzazione dei vertici gestionali. In secondo luogo, per nostro conto è opportuno promuovere un'ottimizzazione delle risorse attraverso forme che diano luogo a sinergie, grazie alle quali la circuitazione degli allestimenti scenici e del personale artistico scritturato e tecnico porti effettivamente ad un risparmio di spesa. Si potrebbero ottimizzare le risorse, a nostro avviso, avviando una politica di collaborazioni nelle produzioni che porterebbe a dei risultati positivi in termini di risparmio. La parola d'ordine dovrebbe essere sinergia tra le fondazioni e non compartimenti stagni tra le fondazioni. La previsione di incentivi fiscali dovrebbe rendere più allettante per i privati la partecipazione che sino ad oggi è stata poco incisiva, fatte salve le rare eccezioni. L'impossibilità poi di poter contare su risorse certe e di conoscere a priori la disponibilità, rende infatti difficile una programmazione corretta e un ricorso al credito che oggi è fin troppo oneroso. Queste economie dovrebbero essere reinvestite nel settore a favore dei giovani talenti. Questo Governo che parla tanto di merito dovrebbe avere una maggiore sensibilità verso i giovani talenti musicali e artistici di cui il nostro Paese è pieno,

A tal proposito, mi preme porre l'attenzione su quella che è una vera e propria questione giovanile che rappresenta una piaga in questo settore. Colgo l'occasione per invitare tutti ad una profonda riflessione sul tema: in particolare, sulla necessità di dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 di cui ho parlato nel mio precedente intervento.

un'alta formazione che desse luogo a diplomi con lo stesso valore dei diplomi universitari. Per cui i nostri giovani talenti, musicali o artistici, potuto competere nei concorsi internazionali alla stessa stregua dei loro colleghi stranieri: questo oggi è ancora impossibile perché non c'è stata un'equiparazione e non sono stati emanati i regolamenti attuativi. Questa è una colpa grave nei confronti dei giovani, soprattutto dei giovani musicisti, attori e talenti nazionali che lasciamo penzolare in attesa di dare corpo ad una riforma già varata. È una responsabilità che pesa sulla gestione del Ministero dell'istruzione e dell'università,

provvedere. Le proposte che il nostro Gruppo ha presentato non intendevano certo voler conservare privilegi, ma soprattutto evitare che fossero i lavoratori a pagare per impostazioni organizzative e scelte gestionali che sono state fallimentari e che naturalmente non possiamo più tollerare. La razionalizzazione e la responsabilizzazione della gestione, l'avvio di sinergie tra le fondazioni, il coinvolgimento di tutti gli enti, la partecipazione dei privati, le economie di spesa anche attraverso l'avvio di forme di collaborazioni tra produzioni: queste erano le linee guida che abbiamo sottoscritto e attraverso le quali si sono sviluppate le nostre proposte emendative, che naturalmente non sono state quasi mai approvate, tranne felici eccezioni, tant'è vero che alcune di esse sono state accolte. Lo stesso ministro Bondi - che naturalmente continua a non ascoltare - ha sottolineato la necessità di avviare strategie sinergiche tra fondazioni e cooperazioni tra produzioni: non possiamo quindi che rammaricarci del fatto che proposte che andavano in questo senso non siano state sottoscritte, né votate. A nostro avviso, l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo per mantenere in vita il settore, la previsione di strumenti di raccordo tra i diversi enti, la destinazione di una quota crescente di stanziamenti in base alla qualità (perché questo è importante), l'incentivazione di un adeguato sostegno economico da parte dei privati, l'incremento della produttività e la garanzia di una maggiore stabilità del settore, nonché una chiara definizione della responsabilità della gestione all'interno dei vari statuti dovevano essere le linee guida che avrebbero dovuto accompagnare un'organica riforma del settore. Al contrario, mi dispiace dirlo, si è preferito optare per un intervento parziale. Caro Ministro, siamo andati indietro con il passo del gambero: l'intervento è poco incisivo, fatta eccezione per le ripercussioni negative che si manifestano ai danni dei lavoratori del settore. Sotto il profilo spinoso della contrattazione non possiamo che augurarci che si possa addivenire quanto prima alla stipula del contratto nazionale di lavoro e che in questa sede sia possibile legare la contrattazione integrativa all'effettiva produttività. Là dove i conti lo permettano, siamo altrettanto convinti che debba essere realizzato un *turnover,* per non penalizzare solo ed esclusivamente le maestranze. Sarebbe disonesto non riconoscere che alcuni passi avanti anche con questo decreto sono stati compiuti. tuttavia gravi le prese di posizione di questo Governo nei confronti della cultura; la marcia indietro del ministro Tremonti in merito alla lista di proscrizione contenuta nella manovra economica lo testimonia ampiamente. Più volte il Capo dello Stato, non ultimo in questa occasione, al momento della firma del decreto al nostro esame, ha ritenuto di dover intervenire a salvaguardia della cultura; la sua sottoscrizione di questo provvedimento è stata subordinata alla disponibilità all'ascolto da parte del Ministro delle problematiche sollevate dal comparto e dalle stesse opposizioni. Siamo profondamente coscienti delle difficoltà di questo momento e ne sentiamo anche la responsabilità e tutto tutto questo non ci permette di essere più tolleranti nei confronti di gestioni disinvolte e irresponsabili, nei confronti soprattutto degli sperperi; fa parte della nostra cultura, Ministro. Ottimizzare e razionalizzare l'organizzazione e la gestione devono essere effettivamente le priorità cui puntare; la forma e la dimensione dell'intervento devono essere necessariamente rispettose della dimensione culturale, che è l'identità di un popolo e ne determina profondamente il suo progresso o la sua drammatica involuzione: e questo, signor Ministro, lei lo sa bene e lo testimonia spesso anche nei suoi discorsi. In tal senso, auspichiamo quindi che gli interventi in materia culturale non siano più considerati alla stregua di spese inutili, ma vengano considerati come investimenti. Un Paese che non investe nella cultura, nell'arte, nella musica, nello spettacolo e nel cinema è un Paese che taglia i ponti con il suo futuro e con quello delle sue giovani generazioni, che ne mortifica la creatività, l'unico valore aggiunto che possiamo dare alla nostra economia a costo zero. zero. Dobbiamo puntare sulla cultura, sulla creatività, sui talenti, perché questo Paese risorga sotto il profilo di una dignità culturale che sta perdendo giorno per giorno e risorga soprattutto nelle aspettative dei giovani e della loro dignità a costruirsi un futuro secondo il proprio progetto di vita e le proprie vocazioni individuali. Se mortifichiamo e continuiamo a mortificare le loro coscienze, la loro intelligenza e le loro capacità non daremo nessun futuro alla nostra democrazia. Si abbia quindi il coraggio di essere effettivamente più fedeli alla nostra identità nazionale che sta nella nostra cultura.

uno spazio dignitoso nell'ambito della globalizzazione di cui tutti parlano. Se continueremo di questo passo anche coloro che venivano dalla Corea o da altri Stati dell'Est a studiare nei nostri conservatori, a vivere la vita dei nostri teatri non verranno più.

che ha sempre illuminato lo spazio dell'arte in Italia, in tutti i suoi campi. Per queste ragioni, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario a questo provvedimento e si augura che il Governo sappia in futuro fare meglio. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'approvazione dell'emendamento 1.100 da noi presentato a questo decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche riafferma, in parte, i principi sottoscritti all'unanimità nella risoluzione votata nella 7a Commissione il 18 marzo 2009, della quale sono stato uno dei due relatori. Anche se il fatto che talune disposizioni siano state espunte in quanto presentano difficoltà di ordine finanziario, non ci consente di dichiararci del tutto soddisfatti,

cui si è successivamente aggiunta la proposta innovativa di ispirazione federalista della Lega Nord (disegno di legge n. 1422, presentato dal senatore Luciano Cagnin). Evitato il rischio di affrontare frettolosamente l'argomento nell'ambito di questo provvedimento, ci auguriamo che il cinema torni in tempi brevi all'attenzione della 7a Commissione e trovi adeguato consenso la visione più attenta al territorio della Lega Nord. Ma torniamo alle fondazioni. È troppo facile, senatore Casson, proporre dall'opposizione lo stanziamento di risorse per una fondazione sapendo benissimo qual è l'attuale condizione della finanza pubblica. Ci penserà il federalismo a mettere le cose a posto! Quali sono, invece, i principi che hanno trovato spazio nel provvedimento e sui quali contiamo per costruire un diverso futuro del mondo delle fondazioni lirico-sinfoniche? elenco alcuni: prevedere specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; adottare ogni opportuna iniziativa, ove necessario anche a carattere normativo, volta a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse; costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; richiedere alle fondazioni lirico-sinfoniche che gli statuti attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale (ovvero sovrintendente) la responsabilità della gestione che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale; prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa, mantenendo la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo (lirica, balletto, musica sinfonica) come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni; valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali verso cui, del resto, sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali nazionali; prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative. Crediamo siano motivi sufficienti per esprimere come Lega Nord, in un momento difficile per l'economia non solo nazionale, un voto favorevole al provvedimento. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, alcune volte capita che nella vita di ognuno di noi si presentino occasioni che aspettano solo di essere colte. Bene, signor Ministro,

a procedere velocemente, con un *iter* legislativo adeguato, ad una nuova normativa che modificava e rinnovava il quadro di riferimento delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Non so spiegare a me stesso e a quest'Aula cosa sia successo. Probabilmente ha prevalso una logica governativa indirizzata a considerare tutto ciò che è cultura, scuola, università, ricerca come un costo e non come un investimento. Non so se sia una scelta meramente revanchista o più marcatamente ideologica; so solo che è una scelta miope, pericolosa, anche antistorica e, soprattutto, drammaticamente sbagliata. In questo decreto‑legge, che ci chiedete di convertire, non si affrontano i temi reali per risolvere i problemi effettivi che hanno creato le difficoltà nelle quali questi enti si sono trovati successivamente alla riforma del 1996. non si è parlato di responsabilità gestionale, di consigli di amministrazione, di produttività, di coproduzioni, di premialità al merito; di risultati e non si è neanche parlato di autonomia responsabile. Si è andati anche contro una pratica di buon federalismo. Si è chiesto invece di delegare al Governo, delegificando la materia, di provvedere con regolamenti ministeriali senza regole, senza controllo, senza l'intesa con il Parlamento e neanche con le Regioni. Signora Presidente, signor Ministro, non era affatto facile fare peggio di così. Contemporaneamente, si umilia un fiore all'occhiello del nostro Paese, la lirica e la musica sinfonica. Si dà uno schiaffo alle Regioni, determinanti per il futuro delle fondazioni stesse. Si considera il Parlamento marginale su una materia che andrebbe modificata con un *iter* legislativo normale e non con un processo regolamentare, inventato nelle ore che hanno preceduto la presentazione del provvedimento. L'interesse del Paese e la politica abdicano nella modesta logica di parte. L'agnello sacrificale lo si è individuato nelle maestranze, negli orchestrali, negli artisti, nei lavoratori tutti delle fondazioni. Si è intervenuti in palese contrasto costituzionale sui contratti collettivi nazionali e sui contratti integrativi; si sono creati dei meccanismi ricattatori, violenti e intimidatori. Si è voluto anche decidere chi tratta per conto di altri ed i tempi nei quali ciò debba accadere, a prescindere, senza mai aprire un serio confronto, senza cercare il consenso delle parti, senza affrontare i temi veri, mai, affossando gli emendamenti che provavano a dare un senso a questo provvedimento. Ma torniamo allo specifico. Ci sono due questioni che si impongono prima di ogni altro elemento nella valutazione del decreto‑legge in questione. La prima attiene ai molteplici profili di legittimità del testo proprio per quanto concerne l'ingerenza sulla contrattazione collettiva; lo hanno ricordato i colleghi Rusconi e Vita nel corso dei loro interventi. Il taglio di una parte della retribuzione integrativa operato mediante decreto-legge è una disposizione senza precedenti. In secondo luogo, la previsione che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico‑sinfoniche sia sottoscritto da una delegazione datoriale, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN e poi sottoposto al controllo della Corte dei conti, appare del tutto incongrua dato che non ci si trova di fronte ad enti pubblici. La seconda questione sulla quale convengono tanti colleghi parlamentari (in sincerità credo anche della maggioranza) attiene alla decisione di procedere per decreto e non attraverso un ben più opportuno disegno di legge. state innumerevoli nei mesi scorsi le promesse del ministro Bondi e del sottosegretario Giro circa la necessità di presentare un disegno di legge e di avviare un'ampia consultazione con gli operatori, con i sindacati, con gli enti locali, con il Parlamento. Nel marzo 2009 all'unanimità la 7a Commissione aveva approvato una risoluzione in cui si invitava il Governo ad aumentare le risorse del FUS, a favorire una maggiore stabilità del settore tramite gli strumenti di finanziamento a carattere pluriennale, a disciplinare con chiarezza negli statuti i compiti dei vari organi, attribuendo - lo sottolineo - la responsabilità della gestione all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, in sintonia con le linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione. Impegni che sono rimasti totalmente inascoltati, perché si è scelta ancora una volta la strada della decisione di imperio. A cominciare dalla presunta urgenza, che giustificherebbe l'uso stesso del decreto, badi bene, per non risolvere i problemi dei maggiori teatri italiani; anche se gli effetti vedranno forse la luce tra 18 mesi. Decisione che non si è piegata neanche alle raccomandazioni del presidente Napolitano, il quale, nel firmare il 28 aprile scorso il decreto, aveva preso atto dell'impegno del Ministro ad incontrare sollecitamente le organizzazioni sindacali ed a prestare la massima attenzione alle preoccupazioni emerse e alle proposte dei Gruppi parlamentari. Eppure noi abbiamo mantenuto quell'impegno, abbiamo provato a modificare questo decreto oggettivamente con grandi difficoltà. Lo abbiamo fatto tenendo conto delle audizioni che si sono susseguite in 7a Commissione: abbiamo ascoltato i sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i sindaci, importanti direttori d'orchestra, i rappresentanti dei lavoratori. Un coro unanime di proteste, di proposte di correzioni significative che sono in gran parte rimaste inevase. Anche recentemente il ministro Bondi ha detto alle agenzie di stampa che il decreto serve per evitare il fallimento del settore. Signor Ministro, mi dispiace, ma ha torto. In questo modo si condanna la quasi totalità dei nostri teatri al declassamento e forse anche alla chiusura. Badate bene, nessuno di noi minimizza i problemi di deficit che riguardano le fondazioni, tantomeno posso minimizzarli io che, come Sottosegretario del Governo Prodi, tante volte mi sono confrontato con tali questioni. Per questo risulta incomprensibile la decisione del Governo di votare contro, di respingere i due emendamenti da me presentati in Aula, che miravano ad introdurre la defiscalizzazione dei contributi delle imprese e dei privati. Il paradosso è che da una parte il Governo chiude il rubinetto dei finanziamenti pubblici e, dall'altra, impedisce di fatto la contribuzione delle imprese e dei privati. Eppure, il Ministro già una volta si era dovuto ricredere sui benefici effetti della *tax credit* sul cinema. Una misura introdotta dall'allora ministro Rutelli, soppressa e poi prevista nuovamente dal Governo in carica. Basta leggere i bilanci delle fondazioni per capire che uno dei nodi irrisolti è la scarsa partecipazione dei privati. Era questo il senso vero delle fondazioni ovvero uno strumento idoneo per attirare capitali privati oltre che il sostegno delle amministrazioni locali, fermo restando un centrale coinvolgimento statale. Se c'è qualcosa che non ha funzionato nella riforma del '96 è stato proprio non prevedere meccanismi consistenti di incentivi fiscali e chiare responsabilità amministrative. Era questo il momento giusto per rivederli, ma il tempo ristretto a disposizione per il dibattito connesso alla decretazione d'urgenza non consente un approfondimento su tali nodi cruciali. Ecco perché non si può certo definire riforma questo testo, ma una messa in mora di un settore culturale così importante per il Paese e per la sua immagine internazionale. Eppure ne esistevano di percorsi alternativi, signor Ministro. Basti pensare al disegno di legge n. 1256, presentato nella scorsa legislatura dall'allora senatore Fontana, che introduceva criteri di premialità rispetto al merito e che maggioranza e opposizione decisero congiuntamente di firmare. Per questo, con la finanziaria 2008 era stato approvato un fondo triennale per la ricapitalizzazione delle fondazioni sulla base di criteri di merito, in ossequio ad una scelta che considero ancora lungimirante. Presidente - insieme a tutta l'opposizione aveva ottenuto alcuni miglioramenti al testo: lo stralcio dell'articolo 5 sul cinema, vista la totale estraneità al testo, ma anche la riduzione dal 50 al 5 per cento della penalizzazione sui contratti integrativi in caso di mancata firma del contratto nazionale. Su questo Governo e maggioranza

così come è successo sull'innalzamento al 30 per cento per le assunzioni a tempo determinato. Quello che di buono - ahimè abbastanza poco - si era riusciti a fare insieme in Commissione, il Governo e la maggioranza qui lo hanno annullato,

Il Partito Democratico voterà contro questo disegno di legge, così come continuerà ad opporsi alla politica di distruzione della cultura italiana.

Nel dibattito in Commissione ed in Aula, l'opposizione si è voluta presentare all'opinione pubblica come unica paladina della cultura nel nostro Paese ed ha tentato di rovesciare sul Governo e sul centrodestra l'immagine di oi barbaroi, un tentativo francamente un po' arrogante, di bassa propaganda, che non ha giustificazione. L'opera lirica e la musica sinfonica - lo ribadiamo senza esibire alcun distintivo all'occhiello - sono ricchezze culturali di grandissimo pregio, componenti essenziali del patrimonio identitario del nostro Paese: rappresentano al meglio il *made in Italy* ed hanno grande rilevanza anche per il turismo culturale. La creazione di questi prodotti culturali di alto pregio è opera meritoria delle fondazioni lirico-sinfoniche; ad esse è affidata la vitale funzione storica di tramandare le nostre straordinarie tradizioni musicali e di balletto. Queste convinzioni, profondamente vissute, sono alla base della preoccupazione del Governo per il grave stato di crisi del settore. Il ministro Bondi ce ne è venuto a parlare in Commissione in ben quattro occasioni, tutte audizioni il 12 novembre 2008, l'11 febbraio 2009 e, quest'anno, il 13 gennaio ed il 3 febbraio. Non capita quasi mai che un Ministro mostri una simile disponibilità nei confronti del Parlamento, non è servito a molto, dato il trattamento che abbiamo subito anche oggi su questo provvedimento. Di questa crisi del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche il Ministro ha fatto una lucida diagnosi: il sostanziale fallimento del decreto legislativo n. 367 del 1996 di trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, a causa del modesto afflusso di investitori privati; il sempre più grave sbilancio tra costi e ricavi per molte fondazioni; gestioni non sufficientemente improntate a spirito di imprenditorialità, efficienza e rispetto dei vincoli di bilancio; il fenomeno deprecabile della frammentazione della contrattazione collettiva in contratti integrativi, responsabili di rilevanti e ingiustificati aumenti dei costi; esigui ricavi dalla vendita dei biglietti; quantità di produzioni annuali di opere liriche, concerti e balletti molto inferiore alla media dei teatri d'opera europei; una produttività complessiva spesso (non sempre) molto inferiore a quella media europea. I dati dei costi e dei ricavi, che qui non ripeto, evidenziano la crisi in tutta la sua gravità, in particolare per alcune fondazioni. Gravità che, come sappiamo bene dalla scienza economica, tende rapidamente con il tempo ad accelerare, divenendo drammatica: *motus in fine velocior*. Di qui la necessità urgente dell'intervento tramite decreto-legge, modalità legislativa divenuta ora assolutamente indispensabile; dispiace che l'opposizione non l'abbia affatto compreso. I tempi per l'approvazione di un disegno di legge sono ormai, nei casi più favorevoli, dell'ordine di un anno e, sopratutto, non sono mai certi. Potevamo attendere un anno? Certamente no: per varie fondazioni l'attesa di un anno sarebbe stata fatale. Desideriamo dare atto al ministro Bondi, oltre che della lucidità della diagnosi, del coraggio delle decisioni prese nel decreto-legge. È atto di coraggio l'assunzione da parte del Governo all'articolo 1 della responsabilità della revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. In questa revisione, che sarà attuata mediante regolamenti ministeriali, si farà in modo di promuovere al massimo efficienza, corretta gestione, imprenditorialità, salvaguardando l'autonomia statutaria di ciascuna fondazione. C'è piena fiducia che una migliore attenzione da parte dei sovrintendenti alle esigenze della buona amministrazione porti al risanamento dei bilanci. Nel 2008 sono state cinque le fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio in rosso: le fondazioni del Teatro comunale di Bologna, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro La Fenice di Venezia, che hanno presentato un deficit complessivo di bilancio di poco più di 32 milioni di euro. Ma già nei preconsuntivi dell'anno 2009 il risultato di bilancio è notevolmente migliorato. È ancora atto di coraggio avere preso di petto nel decreto-legge la questione del contratto nazionale collettivo di lavoro non più stipulato dal 2003, che diventerà la norma contrattuale fondamentale per le fondazioni. Per questo contratto nazionale collettivo nella delegazione datoriale vi sarà una adeguata rappresentanza del MIBAC, coadiuvata da ARAN e Corte dei conti. Ciò in linea con la grande prevalenza nei bilanci delle fondazioni dei contributi pubblici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Contestualmente andrà molto ridotta la rilevanza dei contratti integrativi, che sono stati veri e propri motori di dissesto. Un esplicito apprezzamento meritano anche due altre serie di disposizioni del provvedimento al nostro esame: quelle relative alle nuove età di pensionamento dei ballerini e delle ballerine, entrambe diminuite rispetto a quelle attualmente vigenti, e quelle relative all'avviamento della nuova IMAIE (Istituto mutualistico autori interpreti esecutori), a cui vengono assicurate regole che ne garantiranno il buon funzionamento.

e 23 commi abbiamo dovuto esaminare ben 480 emendamenti, impegnando un tempo di oltre 31 ore; un tempo assolutamente eccessivo. Per riuscire a concludere l'esame del provvedimento in Commissione con il mandato al relatore siamo stati costretti a ritardare l'esame di importanti atti di Governo nonché l'esame di altri disegni di legge. A mio avviso, occorre provvedere urgentemente ad una modifica delle norme del Regolamento che disciplinano l'attività in Commissione che impedisca usi distorti del prezioso tempo in quella sede. Rinnovo la convinta dichiarazione di voto favorevole a nome del Popolo della Libertà.

Giai. Dichiaro aperta la votazione.

Signora Presidente, come è stato già richiamato, noi dobbiamo convertire in legge il decreto-legge n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero*** Io cercherò di essere il più breve possibile, anche per recuperare quel tempo che l'Aula ha in qualche modo dovuto impiegare per il precedente provvedimento (parlo per quel che mi riguarda). Cerco di fare il punto della situazione, partendo dal fatto che la Corte di Cassazione, con la cosiddetta sentenza Ferrini del 2004, ha escluso che la Germania potesse invocare l'immunità dalla giurisdizione per le deportazioni compiute in Italia dopo l'8 settembre del 1943. Successivamente, la Corte d'appello di Firenze ha disposto l'iscrizione di ipoteca giudiziale su Villa Vigoni, un bene dello Stato tedesco adibito ad attività culturale. L'opposizione della Germania verso il decreto di esecutività è stata respinta dalla Corte d'appello. Il 23 dicembre del 2008 la Germania ha iniziato un procedimento contro l'Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, asserendo che il nostro Paese avrebbe violato la norma sulla immunità dalla giurisdizione. Il provvedimento è ancora in corso. Questa è una premessa per poter comprendere i motivi per cui il Governo ha adottato il decreto di cui stiamo oggi discutendo. Con questo provvedimento il Governo ha inteso intervenire su due questioni diverse: la prima riguarda le conseguenze sui rapporti bilaterali tra Italia e Germania di delicate azioni giudiziarie in corso; attiene alla scadenza degli organismi rappresentativi italiani all'estero - i COMITES e i CGIE - che, come noto, sono oggetto di iniziative legislative volte ad un loro complessivo progressivo riordino (iniziative all'esame della nostra Commissione). Venendo al merito, l'articolo 1, al comma 1, dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana. Tale giudizio, come dicevo prima, è ancora in corso, quindi dovremmo avere gli atti finali, e di conseguenza è anche oggetto delle controversie connesse ai titoli esecutivi. Il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa. Il comma 3, infine, reca una norma transitoria, prevedendo l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Benché questa previsione sia formulata in modo generale e astratto, il motivo che ne ha reso necessaria e urgente l'introduzione nell'ordinamento italiano è, come accennato, il contenzioso fra Italia e Germania relativo alle domande di risarcimento promosse nei confronti della Repubblica di Germania da cittadini italiani deportati nel corso del secondo conflitto mondiale in quel Paese per essere utilizzati quale manodopera non volontaria al servizio di imprese tedesche. Secondo una oramai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che ledono valori universali del rispetto della dignità umana. In questi casi, dunque, secondo la Cassazione non è invocabile l'immunità giurisdizionale degli Stati prevista dalle norme di diritto internazionale. Sulla base di questa interpretazione, i giudici italiani hanno proceduto in via esecutiva e cautelare a iscrivere ipoteche su alcune proprietà tedesche. Queste pronunce sono state oggetto di un ricorso presentato dalla Germania nei confronti dell'Italia nel 2008 davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

di giustizia dell'Aja. L'articolo 1 del provvedimento in esame mira, come si è accennato, a superare questo contenzioso. Occorre rilevare che la Camera dei deputati ha limitato l'efficacia della norma di cui al primo comma dell'articolo in esame al 31 dicembre 2011. al fine di rendere chiaro che questo intervento normativo serve essenzialmente a risolvere il contenzioso con la Germania cui si è fatto cenno e non invece a introdurre stabilmente nel nostro ordinamento una modifica in materia di immunità degli Stati esteri, che, come è stato rilevato nel corso dei lavori nell'altro ramo del Parlamento, meriterebbe di essere affrontata in modo più sistematico. Dai lavori della Camera risulta infatti che l'Italia non ha ancora sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite che ha disciplinato completamente la materia nel 2004. La Camera dunque, nelle more delle ratifica di tale Convenzione, ha ritenuto inopportuno varare, come invece previsto dal testo originario del decreto, una disposizione che modifichi in modo permanente l'ordinamento in questa delicata materia. La Camera inoltre ha eliminato ogni riferimento alle organizzazioni internazionali, che sono escluse dalla legittimazione ad agire presso la Corte internazionale di giustizia. Il secondo articolo del provvedimento in esame, come si è accennato, dispone un ulteriore rinvio delle elezioni del CGIE e dei COMITES. Queste elezioni erano state, dal decreto-legge n. 207 del 2008, rinviate al 31 dicembre del 2010. In attesa del generale riordino della materia, l'articolo 2 del decreto dispone che queste elezioni vengano ulteriormente prorogate, ma dovranno comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Fino all'insediamento dei nuovi organi restano in carica gli attuali componenti dei COMITES e del CGIE. Occorre in proposito ricordare che anche le precedenti elezioni dei prima dell'effettivo svolgimento nel marzo 2004, erano state prorogate da tre successivi decreti-legge (il n. 411 del 2001, il n. 52 del 2003 e il n. 272 del 2003).

finestra") *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, come si desume dal titolo stesso, contiene due disposizioni estremamente distanti tra di loro. La norma di cui all'articolo 1 concerne, infatti, la sospensione dei titoli esecutivi nei confronti degli Stati esteri nel caso in cui sia pendente un ricorso presso la Corte internazionale di giustizia in tema di accertamento dell'immunità giurisdizionale. Ove la Corte dell'Aja ammettesse la sussistenza dell'immunità verrebbero infatti meno i presupposti per la validità dei titoli esecutivi. del decreto-legge prevede, invece, un ulteriore rinvio delle elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Si comprende, quindi, come manchi quella omogeneità che dovrebbe caratterizzare le norme aventi forza di legge, così come indicato dalla legge n. 400 del 1988. Già per questa ragione il decreto appare uno dei soliti pasticciacci *omnibus* che questa legislatura ha il primato di aver varato nel maggior numero. Ma non basta: il decreto manca anche dei presupposti che distinguono lo strumento normativo scelto, ossia la straordinaria necessità ed urgenza del decreto legge, così come sancito dalla Costituzione. Sebbene taciuti nella legge e nella relazione illustrativa, infatti, sia il primo articolo che il secondo sono volti a risolvere dei problemi concreti: per il primo articolo la questione è rappresentata dal contenzioso italo-tedesco sulle richieste di risarcimento presentate dalle vittime della deportazione nazista, le quali, divenute esecutive in seguito a varie pronunce delle corti italiane, sarebbero state impugnate dalla Germania con un ricorso alla Corte internazionale di giustizia nel 2008. Il secondo articolo cerca invece di sanare il ritardo con il quale si sta procedendo alla riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Questioni concrete che il Governo avrebbe potuto risolvere utilizzando, invece che la sua potestà normativa, gli strumenti diplomatici e politici. Infatti l'urgenza che il Governo invoca, e cioè il ricorso presentato dalla Germania alla Corte internazionale di giustizia, così come la scadenza della prima proroga nell'elezione dei COMITES, che era stata fissata al 31 dicembre 2010 senza che la riforma sia stata varata, sono in realtà frutto di un totale disinteresse. il ricorso tedesco è stato presentato nel 2008, ma già nel 2004 la Corte di cassazione, così come ricordato dal relatore, si era pronunciata a favore delle vittime del nazismo. Dovevate aspettare proprio il 2010, con l'acqua alla gola, per emanare un decreto legge che bloccasse tutta la procedura delle disposizioni esecutive nei confronti della Germania? Non poteva il Governo attivarsi prima, cercando una soluzione diplomatica e politica di accordo con la Germania? Non poteva in alternativa procedere con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, che ha disciplinato complessivamente la materia della immunità degli Stati esteri il 2 dicembre del 2004? Doveva proprio operare tramite decreto-legge, lasciando quei cittadini italiani che hanno patito gli orrori del Terzo Reich senza il ristoro morale ed economico che la giurisprudenza aveva loro garantito? Si parla di 200 persone, per le quali attendere un anno o due in più costituisce non solo uno schiaffo simbolico da parte di un Paese come l'Italia che indice il Giorno della memoria ma poi si dimentica dei vivi; ma anche forse, considerando che sono persone di una certa età, questo congelamento dei titoli esecutivi può davvero privare per sempre loro e le famiglie del dovuto risarcimento materiale! Ora, che l'urgenza derivi da un ritardo che ha portato l'Esecutivo con l'acqua alla gola senza adire le vie politiche e diplomatiche ma solo quelle della decretazione d'urgenza, è davvero paradossale. Stesso discorso vale per il secondo articolo: la riforma dei COMITES e del CGIE giace in Commissione esteri al Senato da più di un anno. Adesso allunghiamo i tempi di ulteriori due anni e mezzo: questa la previsione che fa il Governo del tempo che occorrerà al Parlamento per varare la riforma. Anche io ho presentato un disegno di legge che abolisce il CGIE, in quanto ritengo che con l'introduzione dei parlamentari eletti all'estero il Consiglio sia diventato uno strumento di rappresentanza pleonastico ed obsoleto, vittima delle posizioni di potere ed incapace di rispondere al meglio alle problematiche dei nostri concittadini all'estero, cosa che invece riescono a realizzare più incisivamente i COMITES, che sono direttamente elettivi e delocalizzati sul territorio. Ebbene, mi rivolgo al rappresentante del Governo. Se questo Parlamento non fosse intasato a discutere di decreti-legge da voi presentati come se fosse il modo ordinario di legiferare; se le Commissioni non fossero state sfiduciate riducendole a mere sale di attesa dove le leggi di iniziativa parlamentare, soprattutto nel caso di proposte dell'opposizione, attendono di trovare un varco fra quelle di iniziativa dell'Esecutivo; se la Commissione esteri non si stesse riducendo ad un semplice ufficio ratifiche, dove i trattati internazionali vengono approvati senza nulla poter proporre in materia di politica estera, forse la Commissione di cui faccio parte avrebbe avuto i modi ed i tempi per approvarla questa riforma dei COMITES e del CGIE, e i cittadini residenti all'estero non avrebbero dovuto essere privati del diritto di voto nella scelta dei propri rappresentanti, con un ulteriore posponimento che va a mantenere negli organi rappresentativi gli stessi soggetti, per di per di più su base totalmente volontaria, per ben nove anni. In pratica, se ne delegittima l'operato e si svilisce ancora di più la nostra politica in materia di italiani all'estero. Prima i tagli agli istituti di cultura, poi le riduzioni per i corsi di lingua e l'assistenza sanitaria, quindi la soppressione di alcune sedi consolari, infine il congelamento degli organi rappresentativi. I nostri italiani nel mondo, una risorsa culturale ed economica preziosissima, che non solo costituisce un'appendice del nostro Paese ma opera anche da ambasciatore informale dell'Italia nel mondo, mai sono stati tanto bistrattati come da questo Governo. Cari colleghi, questo decreto-legge nuoce a tutti e con le pezze che prova a mettere all'ultimo minuto non accontenta nessuno: non i giudici della Corte di cassazione che con la sentenza del 2004 hanno varato un principio importantissimo per il quale il diritto umanitario è sovraordinato alle norme internazionali in materia di giurisdizione degli Stati esteri; non le vittime della deportazione, civili e militari; non i cittadini italiani all'estero. Verrebbe da chiedere: La superficialità estrema del Governo è ciò che contestiamo: la mancanza di dibattito parlamentare ha impedito di trovare alternative nella soluzione del contenzioso italo-tedesco, ma il decreto reca anche il rischio che questa norma apra un precedente per il quale qualsiasi altro Stato potrà presentare ricorso alla Corte internazionale per bloccare i propri obblighi verso un altro Stato. Come Italia dei Valori abbiamo presentato un emendamento per sanare il secondo articolo del decreto, chiedendo che al rinnovo dei COMITES si addivenga entro il 30 giugno 2011, ma francamente ritengo la prima parte del decreto inemendabile. Attendiamo di sapere se almeno sul secondo punto questo Governo, responsabilmente, vorrà ridurre il vuoto rappresentativo che si creerebbe con il decreto licenziato dalla Camera, anche per valutare che tipo di voto esprimere come Gruppo.

mi obbliga a chiarire ed utilizzare questo tempo di discussione generale per fare luce su questo provvedimento, a chiarire anzi a strachiarire, onde evitare che vi sia ulteriore confusione e che nascano inutili equivoci. Posso anche capire evidentemente il ruolo dell'opposizione, però, non posso accettare che che le verità vengano manipolate.

per esaminare il primo articolo, che riguarda proprio il principio del diritto internazionale e dell'immunità degli Stati dalle giurisdizioni. Ovviamente in questo caso si parla della giurisdizione italiana. Quindi, esiste un principio di diritto internazionale riconosciuto a livello planetario del quale evidentemente l'Italia non può non prendere atto,

a fronte della tutela di questo principio, si decide, evidentemente con necessità ed urgenza, di sospendere fino al 31 dicembre 2011 l'efficacia dei titoli esecutivi nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi la Corte internazionale di giustizia. è stato inserito questo termine, quindi una ghigliottina al 31 dicembre 2011, ed è stato votato un ordine del giorno che impegna il Governo a tenere presente di dover risolvere l'annosa questione di riconoscere anche all'interno delle nostre norme il principio suddetto.

emerge la problematica dei risarcimenti. Come detto prima, nessuno intende mettere la testa sotto la sabbia e per questo sia la Lega Nord, con un ordine del giorno presentato in Aula, sia il relatore, senatore Tofani,

a risolvere l'annosa questione dei risarcimenti nei confronti delle vittime italiane del nazismo. Il tutto, però, deve avvenire, evidentemente, attraverso canali diplomatici in modo da poter risolvere quanto prima l'annosa questione. Ebbene, se il Governo accetterà questo impegno, tale fatto già demolisce tutte le critiche che che il collega Pedica poc'anzi ha elencato perché palesa una volontà, da parte sia di questa maggioranza sia del Governo, di riconoscere certamente un diritto internazionale del quale non si poteva non riconoscerne l'esistenza, ma anche la volontà di impegnarsi a risolvere il problema che emerge dal riconoscimento di questo diritto.

si è a conoscenza che già nell'ultima assemblea del CGIE è stata contestata la prima proroga al 31 dicembre 2010, ma sappiamo anche che proprio ora al Senato è in esame la legge che riforma proprio la materia riguardante i Comites, il CGIE e le modalità di voto. Quindi, se si votasse oggi vi sarebbe il rischio,

quindi emerge la necessità e l'urgenza di rinviare queste elezioni al 31 dicembre 2012, termine questo che dovrebbe tenere conto dei tempi d'approvazione del testo unificato riguardante la riforma degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero,

è stata prevista la possibilità di andare alle votazioni degli organismi in oggetto «immediatamente dopo l'entrata in vigore della riforma attualmente in esame al Senato». Quindi, se la lingua italiana è ancora abbastanza chiara, credo che una dicitura di questo tipo non possa lasciare dubbi sulla buona volontà e sulla correttezza, sia della maggioranza che del Governo.

la conversione in legge del decreto-legge per l'ulteriore rinvio delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che arriva in quest'Aula dopo l'approvazione della Camera dei deputati, presenta alcuni di quegli aspetti di forzatura, di insensibilità e di illogicità che hanno caratterizzato da un paio di anni a questa parte le politiche governative per gli italiani all'estero. Il rinvio del rinnovo dei due organismi elettivi in questione ci viene presentato oggi in appena uno dei due semplici articoli del decreto-legge in discussione, dopo essere stato accorpato nel testo del decreto, con discutibile logica e appropriatezza, alle disposizioni di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana: due temi ben distinti, lontanissimi per loro natura e portata l'uno dall'altro, la cui confusa e precipitosa unificazione tradisce la ormai ben nota volontà di qualche insofferente membro dell'Esecutivo - o dell'Esecutivo nella sua collegialità di sminuire l'incidenza della forte e attiva presenza degli italiani all'estero e delegittimarne gli istituti di rappresentanza elettiva. Per prima cosa non esiste assolutamente quella straordinaria necessità ed urgenza che si attribuisce al provvedimento, dal momento che una riforma per certi aspetti sostanziali dei COMITES ebbe luogo nel non lontano 2003. In secondo luogo (e questo è ancora più importante, inquietante e anche offensivo per gli italiani all'estero), si tratta di un secondo rinvio portato fino a dicembre 2012, che verrebbe ad allungare, stiracchiare di tre anni la durata di Comites e come per attendere la morte per inerzia dei due organismi, la cui scadenza è stabilita su base quinquennale dalla legge istitutiva. Dovevano essere rinnovati nel 2009, ne fu decretato il prolungamento al 2010, e magari fino a quel punto la situazione poteva sembrare tollerabile, ma ora spingere fino alla fine del 2012 è francamente, come ho già detto, una forzatura del tutto ingiustificabile e inaccettabile. Mi domando: i componenti di quale altro organismo istituzionale tollererebbero prima la proroga di un anno e, subito dopo, a tamburo battente, un'altra proroga di due anni, perché nel frattempo se ne contempla, magari, un graduale smantellamento? Infatti, la deliberazione del Consiglio dei Ministri si appella ipocritamente alla necessità di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero. il disegno di legge di riforma di COMITES e CGIE nella cosiddetta bozza Tofani è fermo, parcheggiato, arenato in Commissione affari esteri, e nessuno in possesso di un minimo dì buon senso può venirci a dire che ci vorranno altri due anni per licenziarlo in Commissione e portarlo nell'Aula del Senato per poi proseguire l'*iter* - che potrà essere ancora più difficile e contrastato - nell'altra Camera. Tutti, indistintamente, inequivocabilmente, all'unanimità, i componenti dei COMITES e del CGIE sparsi nel mondo, chiedono a gran voce direttamente e attraverso le conferenze continentali, attraverso l'assemblea plenaria e attraverso il comitato di presidenza del CGIE, che si vada subito, a legislazione vigente, al rinnovo dei due organismi istituzionali, Comites e CGIE e si ponga fine ad una indecorosa farsa che sta trascinando fino al ridicolo e all'insostenibilità quelle che dovevano e dovrebbero continuare ad essere le democratiche rappresentanze elettive di base degli italiani all'estero. Semplicemente avere avuto la sfrontatezza e l'impudenza di prorogare non di uno, ma ora fino a tre anni COMITES e CGIE costituisce un insulto ai cittadini residenti al di fuori del territorio nazionale, in massima parte in Paesi a conduzione democratica, dove decisioni politiche, come questo irragionevole stiracchiamento dei termini di organismi istituzionali non sono neppure immaginabili. Trattare in questo modo quattro milioni di elettori italiani all'estero, l'equivalente di una regione italiana di medie proporzioni, e le decine di milioni di oriundi è un'indegnità per un Paese di emigrazione e di immigrazione. ai senatori della maggioranza eletti all'estero, se ce ne sono questa sera in Aula, perché convincano quanti più colleghi possibile della loro parte a far decadere questo illogico decreto a respingere questa ulteriore offesa ai nostri connazionali nel mondo. Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà favorevolmente

lo abbia detto con il suo prescritto pronunciamento la Commissione affari costituzionali, il che pure ha il suo valore, ma perché così è nei fatti. La requisitoria che abbiamo adesso ascoltato relativamente alla proroga in materia di COMITES e CGIE è assolutamente infondata e pretestuosa; e pretestuosa; replicherà sicuramente per noi il senatore Tofani, relatore, ma direi anche che la risposta è già nel testo dell'ordine del giorno che egli stesso si è dato carico di redigere e sul quale saremo chiamati a pronunciarci con il voto. Il tempo è pochissimo ed è inutile ripercorrerne i passaggi, ma è eloquentissimo; se si è d'accordo sul contenuto di quell'ordine del giorno si vede che sono pretestuose le polemiche. D'altro canto, è altrettanto vero, e tutti lo sappiamo, che sono all'esame provvedimenti, in particolare una proposta che non è di facile soluzione in tutti i suoi passaggi, perché non vi è è totale consenso tra le forze politiche e neppure tra coloro che devono essere i destinatari ed applicatori di queste norme. Con senso di responsabilità, facendoci carico di questo complessissimo problema, si sta proprio esaminando nei tempi adeguati e non incalzanti (come taluni vorrebbero) tutta la materia delle elezioni di questi organismi di rappresentanza democratica dei nostri connazionali all'estero. Per quello che concerne, invece, il primo punto devo solo dire che il Governo ha decretato seguendo una linea di concretezza, di realismo, di buon senso: tre caratteristiche che debbono assolutamente essere conservate in controversie di questo genere. Con metafisica sentenza la Corte di cassazione ha stabilito un principio, sul quale si può ideologicamente discettare fino all'inverosimile, ma che non credo porterebbe grande utilità

Non c'è dubbio che si tratta di una proiezione contenziosa di fatti che ci riportano ai dolori, alle tragedie dell'ultimo conflitto mondiale, ai nostri concittadini deportati in Germania e assoggettati al lavoro forzato, così come - vorrei dire - ci riporta alla memoria di altri numerosissimi nostri concittadini deportati o imprigionati nei campi di concentramento della Russia sovietica, o americani, o inglesi, che hanno dovuto soffrire e patire i lavori forzati in condizioni non dissimili. Ma tutto questo si tramuta in azioni giudiziarie che sono regolate da un contesto, da una cornice internazionale dei rapporti tra gli Stati, che rischia di alimentare attese poi deluse o di essere prese per il verso sbagliato. Noi come Governo, come maggioranza, si è naturalmente solidali con le legittime aspettative dei nostri connazionali che abbiano subito e che, quindi, abbiano legittima aspettativa al risarcimento, ma tutto questo si muove nel realismo, nella concretezza. Attendere che la Corte costituzionale si pronunci, risolva questi delicatissimi nodi dalle implicanze non lievi, che non sfuggono a chiunque abbia senso e responsabilità di Governo; attendere che la Corte si pronunci su questa questione fondamentale di diritto internazionale, mi sembra il minimo che un Governo responsabile possa fare nell'interesse, non solo e non tanto dei rapporti internazionali, ma della tutela delle legittime aspettative dei propri concittadini.

Signora Presidente, innanzitutto vorrei rilevare come ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto‑legge che contiene delle 2. Mi occuperò soltanto dell'articolo 1, perché dell'articolo 2 ha già parlato il collega, senatore L'articolo 1 dispone la sospensione di diritto dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero fino al 31 dicembre 2011, qualora sia pendente dinnanzi alla Corte internazionale di giustizia un ricorso diretto all'accertamento delle immunità

uno Stato estero non potrebbe essere convenuto in giudizio dinnanzi ai nostri tribunali per atti che investono la sua sovranità. Può invece essere convenuto, come è notorio, per atti posti in essere alla stregua di un privato. La distinzione, quindi, di atti *iure imperii* ed atti *iure gestionis* vale, *mutatis mutandis,* anche per i beni che possono essere sottoposti a misure esecutive. è intervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza Ferrini dell'11 marzo 2004, la quale ha escluso che la Germania potesse invocare l'immunità dalla giurisdizione per le deportazioni compiute in Italia dopo l'8 settembre 1943. Quindi, ci si inserisce in un contenzioso ben preciso che è bene che venga ricordato in maniera esplicita. Questo contenzioso traeva origine dalle terribili vicende della Seconda guerra mondiale nell'ambito dei crimini commessi in quel contesto, in violazione del diritto umanitario, da truppe occupanti nei confronti delle popolazioni civili o anche di prigionieri in uniforme. Si trattava di eccidi per rappresaglia contro atti di resistenza, deportazioni forzate e lavoro coatto, nonché di internamenti di militari che perdevano lo *status* di prigionieri di guerra ed erano costretti al lavoro forzato. Ricordo che si trattava di fatti concernenti le truppe tedesche del Terzo Reich che però in futuro potrebbero essere quelle di altri Stati per per atti commessi nello stesso periodo storico in altri Paesi occupati o per altri tempi più recenti. Si tratta comunque di fatti che riguardano l'Italia successivi all'8 settembre 1943. Questa sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione italiana ha suscitato notevoli discussioni; i giuristi si sono divisi su questa materia perché si riteneva, da una parte, di dover sostenere la prevalenza del diritto internazionale e, dall'altra, di dover sostenere la prevalenza del diritto umanitario, proprio perché quantunque si trattasse, nel caso di specie, di atto *iure imperii*, veniva violata una norma imperativa del diritto internazionale, *(ius cogens)*, che ha una valenza superiore rispetto alle semplici norme consuetudinarie. Questa impostazione è stata successivamente confermata con due provvedimenti dalla corte d'appello di Firenze e va ricordato che anche i tribunali della Grecia si sono pronunciati nella stessa maniera. Nel timore che siano adottati in questo periodo storico provvedimenti esecutivi nei confronti di beni tedeschi, a seguito dell'ampio contenzioso sviluppatosi dinanzi ai giudici italiani, il Governo ha predisposto questo decreto‑legge che però non solo pare inidoneo a perseguire le finalità cui è preordinato, ma rischia addirittura di avere effetti pregiudizievoli sul contenzioso riguardante l'Italia. riguardante l'Italia. Questo decreto-legge rappresenta un incentivo per iniziare un giudizio contro l'Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Sarebbe stato allora meglio presentare un decreto‑legge

della Corte internazionale di giustizia o ad una sua sentenza. La strada maestra per lo Stato italiano sarebbe però quella di provvedere rapidamente ad un riordino generale della materia dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione. Esiste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004, aperta alla firma nel 2005, ma che l'Italia non ha ancora firmato, nonostante una serie di Stati europei abbia già provveduto. Questa è la strada maestra per cercare di venire incontro alle esigenze delle vittime delle stragi naziste e anche di armonizzare il nostro ordinamento ai principi del diritto internazionale. Quindi, diamo rapidamente attuazione ed esecuzione alle norme previste da questa Convenzione internazionale!

Presidente, signori senatori, vi annuncio sin da subito che mi asterrò dal votare questo provvedimento, segnatamente in relazione all'articolo 1. lo faccio per ragioni che sono di coerenza rispetto all'atteggiamento della Germania. La Germania, nella sua giurisdizione interna, non molto tempo fa ha elaborato il criterio a tenore del quale, quando sono in discussione valori universali e valori che offendono i principi umanitari, non vale nemmeno, per il diritto penale tedesco, il principio del *nullum crimen sine lege*. I tedeschi sono riusciti a compiere l'orrore di condannare i poveri disgraziati di guardia al confine che, sotto il pericolo di essere immediatamente fucilati, hanno sparato contro quelli che scappavano dalla gloriosa Germania dell'Est.

La sentenza delle Sezioni unite su questo in realtà copia, trasferendolo in tema, un principio che la stessa Germania aveva affermato nel suo ordinamento interno. Ma c'è di più: la Germania, che si appella alla Corte internazionale di giustizia, per quanto attiene alle decisioni della Comunità europea e delle Corti europee,

Chiedo scusa ai colleghi se ruberò ancora qualche minuto, ma mi sembra doveroso per il tema che stiamo affrontando

alla Convenzione di New York del 2004, né alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1972. Quindi, le argomentazioni emerse hanno un significato

Correggere il decreto del Governo e dare una temporaneità allo stesso. Su questa strada noi ci siamo potuti inserire

ponga in essere immediatamente iniziative tali da permetterci di aderire alla Convenzione di New York. Abbiamo avuto rassicurazione da parte del sottosegretario Scotti,

Nello stesso tempo abbiamo cercato di far valere quel concetto fondamentale di carattere umanitario richiamato dal collega Casson.

in questa materia occorre contemperare il rigoroso rispetto delle norme del diritto internazionale generale cui, secondo l'articolo 10 della Costituzione

abbiamo anche voluto specificare che «l'ulteriore rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE è esclusivamente motivato dalla opportunità di completare il procedimento di organica riforma della legislazione

perché non è un tema che spetta al Governo, ma al Parlamento. Ci auguriamo che questo *iter* legislativo possa concludersi, sia al Senato che alla Camera, entro quest'anno,

credo che un Parlamento, di fronte a questi problemi e all'opinione pubblica internazionale, non possa non mostrare

Casson, che sono intervenuti dando un contributo estremamente rilevante alla chiarezza delle questioni da affrontare. Il decreto-legge riveste alle questioni aperte in occasione di provvedimenti esecutivi emessi nei confronti di Stati e di organismi internazionali. Il provvedimento offre soltanto una risposta parziale al problema, perché si riferisce ai procedimenti rispetto ai quali c'è in questo momento un'iniziativa presso la Corte internazionale.

né questo sono arrivati ad una soluzione. Il Parlamento deve trovare una risposta per la complessità delle questioni che sono state trattate e per la divisione che esiste nell'opinione di eminenti giuristi italiani e internazionali. Un'ultima cosa mi sia consentito aggiungere, perché delicata e importante. Accanto a questa azione diplomatica e legislativa c'è un problema: quello di consolidare gesti di peso politico e morale intesi a rafforzare una prospettiva di riconciliazione tra Italia e Germania, segnatamente al livello di società civile, nel segno della comune appartenenza all'Unione europea. In questi ultimi due anni il Governo si è mosso in questa direzione. Sono significative - lo voglio ricordare in questa sede perché resti agli atti del Senato e presente all'opinione pubblica tedesca - la visita alla Risiera di San Sabba da parte dell'allora vice cancelliere, ministro degli esteri tedesco, Steinmeier, il 18 novembre 2008; 2008; l'istituzione di una commissione di storici italiani e tedeschi con il mandato di un approfondimento comune sul passato di guerra italo-tedesco, in particolare sugli internati militari italiani, come contributo alla costruzione di una comune cultura della memoria; memoria; l'avvio presso il Centro italo-tedesco di Villa Vigoni di una piattaforma Internet per lo sviluppo di scambi giovanili tra Italia e Germania indirizzati, in particolare, alla tutela della memoria delle vittime di persecuzioni e stragi naziste; da ultimo, l'impegno della Germania nella ricostruzione di Onna, uno dei paesi abruzzesi distrutti dal terremoto, teatro nel 1944 di una strage di civili da parte di truppe tedesche. Questi sono i risultati importanti dell'iniziativa politico-diplomatica dell'Italia nel contesto di una questione di estrema delicatezza e sensibilità per l'opinione pubblica e per il Governo tedesco. Detto questo, il Governo

cioè soprattutto l'invito a sottoscrivere rapidamente la Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e a provvedere di fatto a tutelare le vittime degli eccidi nazisti dopo l'8 settembre del 1943.

comitati eletti a suffragio universale, ma formati da persone che fanno volontariato puro e che non costano nulla allo Stato. Non si può pretendere da persone che danno un servizio di volontariato di questo tipo e che sono stati eletti

Perché chiediamo questa certezza? Porto un solo esempio che ho fatto in Commissione affari esteri pochi giorni fa. Noi abbiamo difficoltà con questo Governo e con l'amministrazione del Ministero degli affari esteri; in questi anni abbiamo avuto l'impressione di avere un dialogo autistico: tutte le

ma non hanno mai trovato accoglienza e possibilità di dialogo con l'amministrazione e con il Governo. Si pensa di risolvere i problemi finanziari. Questa settimana il sottosegretario Scotti ci ha detto che una parte dei tagli

che non accetta alcun dialogo sulle proposte di riorganizzazione e di risparmio che noi avanziamo. Abbiamo portato un solo esempio in Commissione esteri: il consolato generale di Zurigo da anni ha

a questo punto chiediamo di votare il nostro emendamento perché non abbiamo un rapporto di fiducia sufficiente.

mobilitate e organizzate con molto sacrificio, anche personale. Ringrazio gli italiani che fanno volontariato in questi comitati e che si sono riuniti

Il 23 aprile scorso, nella riunione n. 90, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia, ha approvato il decreto legge n. 63 che, oltre a contenere disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana, all'articolo 2 contempla lo spostamento al 31 dicembre 2012 del termine ultimo le elezioni dei COMITES e del CGIE. In merito al suddetto articolo 2, un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri cita testualmente: «Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organismi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalità e delle procedure previste dal citato rinnovo dei medesimi Comitati». Quale straordinaria necessità e urgenza ha il Governo a rinviare queste elezioni? I COMITES e il CGIE dovevano essere rinnovati lo scorso anno,

A che gioco stiamo giocando? Non si capisce. Perché non lasciare invariate le cose? Perché non votare nel 2010, visto che gli stanziamenti (pari a 6 milioni di euro) per il rinnovo dei Comitati sono stati già determinati con legge di bilancio per gli esercizi finanziari cui le spese si riferiscono? Che fine faranno questi stanziamenti? Rimarrebbero sicuramente inutilizzati, mentre occorrerebbe disporre nuove risorse finanziarie per l'anno in cui verranno effettivamente svolte le elezioni. Perché tutto questo accanimento nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero? Perché non rispettare il criterio di parità, che la Costituzione italiana sancisce, tra cittadini italiani residenti all'estero e cittadini italiani residenti in patria? A quanto pare non abbiamo gli stessi diritti. Ritornando ai COMITES e al CGIE, vorrei inoltre ricordare che sono oggetto di uno specifico processo di riforma. A tale proposito auspico

Reputo quindi inopportuno l'inserimento dell'articolo 2 all'interno del decreto-legge, non essendo questo lo strumento più adatto per affrontare l'argomento. Ribadisco quindi la mia contrarietà e preannuncio, anche a nome del mio Gruppo,

*(PD)*. Signor Presidente, volevo in primo luogo ringraziare il senatore Tofani perché, anche se le nostre conclusioni possono essere diverse, ha offerto a questa discussione un'interlocuzione seria e un contributo di approfondimento che io ho apprezzato. Alcune delle cose che il senatore Tofani ha detto corrispondono naturalmente al vero: è vero, ad esempio, che nel corso dei lavori parlamentari questo provvedimento è migliorato, sia nei lavori della Camera ma anche gli ordini del giorno che qui sono stati presentati costituiscono un passo in avanti rispetto al punto dal quale eravamo partiti. Spendo poche parole, però, per affrontare quella che credo sia la questione principale, perché

si presenta quasi come una storia del passato - stiamo parlando infatti dei ricorsi fatti da quei pochi sopravvissuti dei campi di sterminio, del lavoro forzato, della deportazione in Germania: quanti possono essere? Poche persone, ormai

la sovranità nazionale e l'affermazione di principi universali costituisce una delle sfide che stanno davanti alla nostra coscienza e anche alla nostra responsabilità politica. Non vorrei che fossero considerate con sufficienza quelle sentenze dei tribunali e poi della Cassazione che hanno preso una decisione certo discutibile, sulla quale ci sono opinioni controverse, ma che in fondo invoca il principio per il quale c'è un limite alla sovranità degli Stati e che è dato dalla violazione di valori generali, di principi universalmente riconosciuti. E' la ricerca di di questo equilibrio che ci si ripropone continuamente come una questione essenziale. Questo è il punto che mi porta ad esprimere una valutazione preoccupata. in una situazione nella quale c'è, da un lato, una ragione politica e la ragione della sovranità e, dall'altro, stanno le vittime; in cui, da un lato, sta il realismo politico delle relazioni internazionali e, dall'altro, stanno i principi generali, noi non riusciamo a costruire un equilibrio nuovo. Questo è un punto che conferma una realtà politica con la quale continuamente ci misuriamo. Posso dire ciò con una certa pretesa di oggettività perché so che non è una questione che riguarda solo una maggioranza, solo una coalizione: è una questione che sta davanti alla politica italiana e alle sue responsabilità, alla sua capacità di interpretare questa questione. lo voglio dire, senatore Tofani, parlo a lei naturalmente per rivolgermi a tutti i colleghi - la forma del decreto non ci ha aiutato. Il ricorso di fronte alla Corte di giustizia dell'Aja da parte del Governo tedesco è del dicembre 2008. Vi era il tempo per muoversi diversamente; lo dico con dolore. Non siamo riusciti neanche a sentire quelle vittime, quelle associazioni che ci hanno scritto per dire le loro ragioni di deportati. Non abbiamo neppure avuto il tempo per una audizione, per dare la soddisfazione a queste persone di essere ascoltate dal Parlamento che decideva sulla loro vita. E' o no un problema, questo, per tutti noi?

che il Senato meriti su questo punto, nel rispetto delle proprie prerogative, una discussione più attenta di quella che rischiamo di fare. Signor Presidente, non devo vedere la partita, ma in ogni caso rinuncio all'intervento poiché quanto avrei dovuto dire si rispecchia nell'ordine del giorno del collega Tofani, ed il nostro Gruppo voterà convintamente a favore.

L'altro argomento riguarda il senatore Legnini, il quale mi ha invitato a studiare il Regolamento del Senato. Ebbene, da tanta fonte io non potevo sottrarmi a questo dovere. che parla sempre senza che gli sfugga mai un sorriso (perché deve aver fatto una convenzione con qualcuno) e parla con una mano in tasca e l'altra no (perché deve puntare l'indice),

si chiude così: infatti, quando gli Uffici le hanno ricordato che esiste una consuetudine, non le hanno evidentemente ricordato che prima ancora c'è il Regolamento, richiesta deve essere presentata prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Allora, il Presidente invita il Senato a votare soltanto dopo che sono trascorsi nel caso concreto, i tempi di sospensione

che otto lavoratori sono saliti questo pomeriggio sul tetto della azienda per esprimere una protesta. Vorrei chiedere alla Presidenza di sottoporre al Ministro del lavoro questo problema affinché venga a riferirci perché non siano stati rispettati gli accordi. È l'ennesimo caso all'interno di una delle zone più produttive d'Italia, la Brianza. Questi otto lavoratori sono in rappresentanza di molti altri.

ha trasferito la sua attività in un'altra zona della Lombardia, ma non sono stati minimamente rispettati gli accordi che erano stati sottoscritti.

in maniera molto chiara, stabilisce che le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente. Quindi, soltanto dopo venti minuti possono essere indette. Lei capisce che in quel caso si sostengono delle tesi non tanto per una questione di interpretazione regolamentare, ma perché l'Aula comunque è un soggetto politico. Pertanto, in quella fase c'era una forma di contraddizione all'interno della Lega e l'opposizione aveva interesse a farla esplodere interpretando il Regolamento in quel modo. L'importante è che gli Uffici abbiano le idee chiare nell'interpretazione del Regolamento. **Sulla crisi dell'azienda

Non sono a conoscenza se i partiti ed i Gruppi politici abbiano già fatto pervenire le rispettive segnalazioni. Sono viceversa a conoscenza del fatto che si continua a morire a causa dell'uranio impoverito e dell'amianto. Quindi, mi appello alla sensibilità della Presidenza, affinché, con l'urgenza che la gravità della situazione impone, voglia attivamente ed efficacemente adoperarsi perché questa Commissione possa iniziare a lavorare già dai primi giorni di luglio. ha sollecitato in maniera formale i Gruppi che ancora non hanno indicato i propri componenti. Volevo informarla che c'è un invito formale del Presidente del Senato.

visto che come componente della Commissione difesa mi sono adoperato per l'istituzione di quella Commissione che ho anche votato, se eventuali reticenze o ritardi immotivati

responsabilità dei gravi ritardi, possa essere ribaltato a danno di chi li ha prodotti. Senatore Scanu, quando il Presidente del Senato fa una notifica per iscritto lei capirà che si rende conto di ciò che fa e, di conseguenza, sa valutare come regolarsi: una cosa è un invito orale, altra cosa un invito per iscritto.

che prevedevano il ricollocamento e il prepensionamento degli operai, ancora oggi in cassa integrazione. In marzo avevo chiesto al ministro Sacconi di impegnarsi per la concessione della cassa integrazione